Onorevoli colleghi, rendo all'Assemblea il triste annuncio della scomparsa del senatore Ignazio Manunza, deceduto improvvisamente il 24 agosto scorso a sessantasei anni. Fortemente impegnato nella realtà politica della Sardegna, il senatore Manunza aveva una lunga carriera politica alle spalle. Già consigliere regionale e sindaco di Oristano, la sua città, dal 1981 al 1984, era stato eletto per la prima volta al Senato nella XIV legislatura

In Senato tutti lo ricordiamo per il tratto mite e discreto e per l'assidua ed esemplare presenza ai lavori parlamentari in Aula e in Commissione. Alla vedova, signora Adriana, ai figli, ai colleghi del Gruppo di appartenenza e del suo partito, agli elettori della Sardegna esprimo il cordoglio mio personale e dell'intera Assemblea. Debbo e voglio poi anche ricordare con dolore e angoscia l'assassinio di suor Leonella Sgorbati e della sua guardia del corpo, uccisi a Mogadiscio in un atto di atroce violenza. La figura umana e morale di suor Leonella emerge in queste ore con sempre maggiore chiarezza. Una persona che aveva dedicato l'intera sua vita all'assistenza ai più bisognosi, al colloquio e alla comprensione degli altri, fino al sacrificio estremo nobilitato dalle ultime parole con le quali ella ha chiesto perdono per i suoi assassini. Ho già avuto modo di esprimere ai familiari e alle consorelle di suor Leonella il più profondo cordoglio mio e di Palazzo Madama. Nel momento in cui sembrano accentuarsi le ragioni di contrapposizione tra le religioni, dobbiamo tutti lavorare affinché la disponibilità al confronto e al dialogo interreligioso che il Pontefice ha voluto ribadire nel suo discorso di domenica scorsa prevalga fra tutti. Invito l'Assemblea ad osservare un momento di raccoglimento.

eletto in Forza Italia per la seconda legislatura, collega caro, persona saggia dai modi e dal temperamento oculato e razionale. Una persona che ci mancherà, che mancherà al suo territorio, alla sua Sardegna, ai suoi amici, ai tanti amici che abbiamo avuto modo di incontrare ad agosto in occasione delle sue esequie. È stata una scomparsa improvvisa. Preferiamo ricordarlo seduto nei nostri banchi - come ella molto opportunamente ha ricordato sempre attento, personaggio della politica locale, ma anche di quella nazionale; attento ai lavori dell'Aula, presente, non soltanto con il corpo, ma con la mente, sempre attento anche alle esigenze della sua Regione. Non dimentico, non possiamo dimenticare, le sue battaglie per il riconoscimento di alcune prerogative e di alcuni diritti della sua terra, la sua Sardegna. dimenticare la sua storia, la sua militanza politica in quel territorio, dove è stato sindaco ed assessore regionale. È stato un uomo di spicco che ha fatto crescere il suo territorio, la sua Isola. Ignazio Manunza è andato via improvvisamente: nessuno di noi lo immaginava. Vogliamo ricordare di lui l'espressione quasi sorniona, ma pacata e saggia di una persona che sapeva

Con questo ci associamo al dolore dei suoi familiari e dei suoi amici e di tutti coloro che hanno creduto nel suo progetto.

abbiamo vissuto in quest'Aula, nella scorsa legislatura, momenti di confronto a volte molto aspro e intenso. Mi accadeva spesso di girarmi alla mia sinistra e di incrociare immediatamente lo sguardo di un collega al quale non si poteva non essere affezionati: Ignazio Manunza. Aveva una disponibilità espressa anche dal tratto somatico, aveva una saggezza che si rinveniva nelle sue parole, che non erano mai parole fuori posto

Lo voglio ricordare così. È una delle persone che quando sono stato male in Aula mi è stata vicina, più di tante altre; voglio ricordare quel sorriso profondo al quale faceva riferimento anche il collega Schifani, il sorriso di un uomo che sa già cosa accadrà domani, perché ha vissuto con profonda passione il suo passato e con grande consapevolezza

Signor Presidente, il Gruppo della Lega Nord si associa al dolore dei familiari per la perdita del collega Manunza.

mondo deve accomunare la politica italiana e unire questo Parlamento. Crediamo che tale preoccupazione dovrà trovare lo spazio politico per una meditazione sul tema della reciprocità: non è possibile che vi sia una mattanza di cristiani in giro per il mondo e che si possa semplicemente invocare il dialogo. Parimenti, signor Presidente, ci consenta di esprimere il rammarico, ed anche il cordoglio ai familiari, per la perdita di Oriana Fallaci.

alcune delle chiacchierate che facemmo allora e ho appreso soltanto da pochi giorni - quand'è accaduto mi trovavo all'estero - della sua morte. Desidero, quindi, anch'io associarmi

Signor Presidente, anche il Gruppo UDC si associa in modo particolare al dolore del Gruppo di Forza Italia e della famiglia per la morte del senatore Manunza. Non ero, purtroppo, tra coloro che avevano avuto la fortuna

Ignazio stava male da molto tempo; spesso, di fronte a certe malattie, è consigliabile ridurre l'impegno politico, ma era tanto l'amore

ruolo e quanto abbia dato con il proprio lavoro e con il proprio esempio Ignazio, che, insieme a me e ad altri parlamentari di Forza Italia, ha voluto aiutare gli amici della Democrazia Cristiana e del Movimento per l'Autonomia ad avere la dignità di Gruppo

mi fa piacere ricordare a quest'Aula che il problema, tra noi e nei confronti della Fallaci, non è condividere le stesse opinioni, ma rispettare le opinioni degli altri. Nel rispetto di un'opinione differente dalla mia, mi inchino ad Oriana Fallaci. una nuova finestra"). Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere della Giunta per il Regolamento espresso nella seduta del 7 giugno 2006 all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Sardegna a seguito del decesso del senatore Ignazio Manunza, ha riscontrato nella seduta odierna che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il predetto senatore è Fedele Sanciu. Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo senatore Fedele Sanciu. Avverto che da oggi decorre nei confronti del nuovo proclamato il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami. Comunico che, in data 15 settembre 2006, è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Vice presidente del Consiglio dei ministri:* «Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA» Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi, ha definito a maggioranza il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 28 settembre. Come già stabilito prima della pausa estiva, riprenderà da oggi l'esame del disegno di legge recante «Sospensione dell'efficacia di disposizioni Nel corso della seduta pomeridiana di domani, mercoledì 20 settembre, sarà sottoposto alla deliberazione dell'Assemblea il parere contrario della 1a Commissione permanente sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge in materia di IVA. Tale votazione prevede la necessaria presenza del numero legale. Nell'ambito della seduta antimeridiana di giovedì 21 settembre sarà esaminata la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in ordine a una richiesta di autorizzazione a procedere. Il calendario della prossima settimana, oltre al seguito degli argomenti non conclusi, prevede la discussione dei disegni di legge, ove conclusi dalle Commissioni competenti, relativi alla ricostituzione delle Commissioni di inchiesta antimafia e sul ciclo dei rifiuti, nonché delle proposte istitutive delle Commissioni monocamerali di inchiesta sugli infortuni sul lavoro e sull'uranio impoverito. Nella seduta antimeridiana di giovedì 28 settembre sarà discusso il bilancio interno del Senato insieme al rendiconto. Infine, per quanto concerne la vicenda Telecom, il Presidente del Consiglio dei ministri ha preannunciato la propria disponibilità a riferire al Parlamento, con modalità ancora da definire, nella giornata di giovedì 28 settembre. La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi martedì prossimo per un adeguamento del calendario. Poiché ci sono state dichiarazioni e interpretazioni su quali modalità, dove e come il 28 settembre il Presidente del Consiglio riferirà sul caso Telecom, io vi comunico - perché per la distanza che c'è abbiamo incaricato il Governo di prendere i contatti portando la richiesta pressante di molti dei Gruppi

Presidente, questo calendario che ci è stato comunicato e che è stato approvato soltanto a maggioranza,

non ha trovato il nostro consenso per una motivazione di carattere squisitamente politico. In questi giorni si è parlato tanto, ed è sotto gli occhi di tutti come la vicenda che ha dato luogo alle dimissioni dell'amministratore delegato della Telecom

dando luogo a una serie di fortissime perplessità sia all'interno dell'opposizione ma notevolmente anche all'interno della stessa maggioranza. Si è parlato tanto dell'esigenza di chiarezza da parte del Presidente del Consiglio su questa vicenda. Una chiarezza che coinvolge la stessa persona del Presidente del Consiglio, non tanto il Governo nella sua azione collegiale e nella sua linea politica, ma come ma come responsabilità personale e politica del professor Prodi.

ingenerosa del Presidente del Consiglio, che dall'estero si è permesso di dare dei pazzi ai componenti di un ramo del Parlamento che chiedevano di essere ascoltati. *(Applausi dal Gruppo Non vogliamo che nella nostra memoria e nella storia di questo Parlamento rimanga questa ferita. Eppure, abbiamo assistito dapprima ad una reazione scomposta da parte del presidente del Consiglio, il quale giorno prima di questa richiesta aveva dichiarato al mondo intero di non conoscere affatto il piano di dismissione della Telecom

noi ci chiedevamo il motivo. Poi, appresa la notizia che il consulente economico dello stesso professor Prodi aveva mandato a Tronchetti Provera ben altro progetto e che su quel progetto non vi era stata condivisione dell'amministratore delegato, abbiamo capito *a posteriori* le motivazioni della rabbia del Presidente del Consiglio in quanto le sue proposte non erano state accolte. Si è voluto prendere da parte del Presidente del Consiglio le distanze da quanto avvenuto e si è sostanzialmente tentato di fare credere al mondo intero che il Presidente del Consiglio sconosceva l'operato del suo consulente economico il quale lavorava a Palazzo Chigi e inviava dei *dossier* su carta intestata di Palazzo Chigi.

Si è detto che il Governo era pronto a riferire sulla vicenda complessiva riguardante una tematica che interessava 90.000 posti di lavoro e un'azienda che fa parte del sistema Italia, Italia, della telecomunicazione, sulla cui efficienza si misura la competitività di un Paese, e ci si è offerta la possibilità di dibattere con dei ministri che venissero a riferire su questo argomento in senso lato. lato. Noi abbiamo chiesto con forza, ma anche con senso di responsabilità, la presenza del Presidente del Consiglio perché quel dibattito offertoci avvenisse in Parlamento alla presenza dello stesso Presidente del Consiglio affinché facesse tra l'altro chiarezza chiarezza sulla sua linea di politica industriale, se è quella del dottor Rovati suo consulente economico o se è un'altra, quella di altri ministri del suo Governo. Ci è stato detto di no, ci sono state frapposte delle resistenze non indifferenti. Ci siamo impegnati in una Conferenza dei Capigruppo che è durata, con una sospensione di alcune ore, ben quattro ore

effettiva opportunità che il Presidente del Consiglio venisse in Parlamento e non lo fuggisse, che non avesse paura del Parlamento perché è la casa degli italiani, italiani, mezz'ora fa il presidente Marini ci ha informato della disponibilità del Presidente del Consiglio di venire, non giovedì sera, premesso che il Presidente del Consiglio atterrerà a Ciampino giovedì alle ore 12, come apprendiamo da notizie ufficiali di stampa,

di ben otto giorni per preparare il suo intervento. Noi siamo pronti a dargli una mano, ma non crediamo che occorrano otto giorni per venire a chiarire qual è la sua posizione su questa vicenda.

ma ci teniamo ad evitare di essere scherniti nei fatti, non soltanto nelle parole. Siamo stati offesi nelle parole con quella spiacevole espressione; adesso veniamo offesi nei fatti

questo nostro pensiero e che rivendichino la presenza del Presidente del Consiglio in entrambi i rami del Parlamento. Evitiamo conflitti tra Camera e Senato. Non è nel nostro costume. Vogliamo allontanare questa ipotesi, anche perché su una vicenda così delicata riteniamo che il Presidente del Consiglio debba informare il Parlamento nella sua interezza e compiutezza. Ecco perché non condividiamo questa proposta di calendario e ci permettiamo di introdurre una variante che preveda la destinazione di una seduta pomeridiana nella giornata di giovedì affinché

Presidente, come abbiamo avuto modo di esprimere già durante la Conferenza dei Capigruppo, noi siamo contrari a questo calendario.

riferito che il Presidente del Consiglio poteva venire a riferire in Parlamento se noi avessimo presentato un'interrogazione per il *question time,* poi nel pomeriggio, quando abbiamo ripreso i nostri lavori, abbiamo saputo che il Presidente del Consiglio si è dichiarato disponibile a venire a riferire il 28 settembre. Evidentemente, quel Presidente del Consiglio, che lontano dall'Italia aveva detto che era da matti chiedere un suo intervento nelle Aule parlamentari, ha bisogno di dieci giorni di tempo per studiare il caso, per preparare il suo intervento e venire a riferire alla Camera o al Senato. Non chiediamo

dopo un'ampia discussione che ha coinvolto anche il Governo, ha deciso di intervenire in Parlamento il prossimo 28 settembre.

credo stiano a zero e non valgano nulla. Qui il tema allude ad un grande problema: un bilancio delle privatizzazioni, la bancarotta del Governo Berlusconi per quanto riguarda la politica economica, l'indirizzo di politica industriale, le tendenze del mercato tecnologico, il governo pubblico delle reti come interesse nazionale del sistema delle telecomunicazioni. Vogliamo discutere dei posti di lavori (ad ottobre vi è un'iniziativa sindacale); vogliamo discutere di quanto compiuto da Francia e Germania anche in termini normativi in Parlamento. I giorni ci servono per questi temi; è di questo che vogliamo discutere, non di *gossip* o di responsabilità individuale del Presidente del Consiglio, ma del fatto che ancora una volta si rischia di perdere l'ultimo settore strategico in cui l'Italia conta qualcosa nella divisione internazionale della produzione dei lavori. Si rischia di perdere, dopo una privatizzazione peraltro sbagliata, un settore importante come quello delle telecomunicazioni. Di questo vogliamo parlare ed infatti abbiamo avanzato,

discutere e affrontare il tema di fondo che è, ripeto, quello della politica industriale, il rapporto pubblico-privato, gli indirizzi che il Governo e il Parlamento possono, nei confronti di una grande azienda di un settore strategico, fornire e ricevere. Di questo vogliamo parlare, non di propaganda, non di *gossip* e di responsabilità di Rovati. il Paese, i lavoratori, le lavoratrici, i sindacati e il Parlamento possano elevarsi a una discussione seria di politica economica. Per questo approveremo il calendario.

Schifani e Matteoli hanno già articolato e argomentato i motivi per i quali non ci siamo sentiti di votare questo calendario. Non tornerò sulle questioni già aperte, ma

delegato Tronchetti Provera illustra un piano di riassetto della Telecom che prevede probabilmente lo *spin-off* i fatti ci dicono che il Presidente Prodi reagisce in maniera stizzita e anche violenta, dicendo che non ne sapeva nulla,

dimette e al suo posto arriva il demiurgo, il *deus ex machina* di questi ultimi tempi delle vicende politiche, economiche e calcistiche italiane, Guido Rossi. Credo che questo sia un tema non di secondaria importanza. Nessuno lo ha mai sollevato, ma credo che dobbiamo domandarci come mai proprio Guido Rossi viene nominato a capo della Telecom. Intanto, devo far rimarcare che non appena la sinistra va al Governo comincia a pasticciare con Telecom. Questo è il punto fondamentale *(Applausi dai non ancora chiariti di Telekom Serbia, quando, guarda caso, proprio Guido Rossi era alla guida di Telecom; accade ancora oggi e ritorna lo stesso personaggio. Ricordo che dagli uffici di Guido Rossi è uscita la prima denuncia sulla questione dei furbetti del quartierino;

che cosa Guido Rossi, Prodi e Tronchetti Provera si sono detti in questi giorni; su questo non c'è il minimo dubbio. Bene, allora dobbiamo interrogarci; io sono inquieto su questo personaggio. Ricordo che la Telecom non è soltanto una delle più grandi aziende italiane, non occupa soltanto uno dei settori strategici nella sfida della globalizzazione: la Telecom è il grande fratello che ci controlla. controlla. Il fatto che da oggi, in qualche modo, ci possa essere Prodi che indirettamente, tramite i suoi sodali, controlla le nostre telefonate non mi lascia assolutamente tranquillo. *(Applausi dai che dobbiamo assolutamente sottolineare. Non è fantascienza, purtroppo, perché abbiamo visto che Telecom, in questi ultimi tempi, è stata protagonista di episodi estremamente oscuri. Mi riferisco alla vicenda Abu Omar, dove ci sono stati anche dei morti legati a queste oscure vicende. Bene, occorre che si faccia chiarezza su questo punto, una chiarezza estrema. Mi stupisce che non sia la maggioranza a pretenderla, quantomeno in Senato. dei Capigruppo è successa una cosa abbastanza strana: abbiamo visto dei Capigruppo della sinistra difendere a spada tratta il fatto che Prodi volesse, bontà sua, rispondere ad un *question time*. Pensate, due minuti;

a dimostrazione della confusione che regna in questo momento nella maggioranza su un tema del genere. Mi dispiace che questo soprassalto di dignità a difesa del Parlamento sia venuto dalla Camera e non dal Senato, che viene quotidianamente calpestato da questo Governo. Ancora una volta c'è il tentativo che in Senato non si discuta. Voglio ricordare che, se Prodi deciderà o se il presidente Marini non sarà in grado - io spero di sì - di difendere le prerogative del Senato, di questa questione il Senato non discuterà, perché evidentemente, per una questione di dignità, non siamo disposti a discuterne - non me ne voglia il ministro Gentiloni - con un Ministro che in questa vicenda c'entra poco o nulla. C'è un'altra questione per la quale non siamo d'accordo su questo calendario; di una questione che intendo sollevare con forza e che solleva la Lega, da sola. Riguarda il silenzio assordante che si è levato in questi giorni, da tutti i Parlamenti europei, sulla vicenda di Benedetto XVI. *(Applausi dai Gruppi* Questo è uno scandalo! Lo scandalo non sta nella violenza del mondo islamico, nel fatto che oggi non è stato più il settore dei terroristi, dei cosiddetti integralisti islamici, a cercare di chiudere la bocca

di Benedetto XVI, ma della libertà. Non ci vogliono più nemmeno far parlare, questo è assolutamente intollerabile! Noi chiediamo che questa mozione venga discussa immediatamente, perché riteniamo che sia la questione più importante che, in questo momento, il Parlamento deve discutere. Non me ne vogliano i magistrati, se magari non vedranno soddisfatta la loro sete di revanscismo e di vendetta contro il provvedimento di riforma dell'ordinamento giudiziario che tanto scandalo ha suscitato. Questa è un'altra questione, che può aspettare anche qualche giorno. Questo è il motivo fondamentale per cui non possiamo approvare questo calendario.

conversando con i nostri colleghi, di sentire espressioni di critica per come i *media* trattano i nostri lavori;

non offrono adeguato risalto alla qualità dei temi che vengono trattati in Aula. Credo che anche

Signor Presidente, ci troviamo davanti alla crisi, molto grave, di un' azienda italiana che svolge un' attività delicata in un settore strategico: un' azienda che da più di cinque anni presenta un indebitamento medio superiore a 40 miliardi di euro

presente questione è sorta dopo una decisione del consiglio d'amministrazione di Telecom assunta una settimana fa che, contraddicendo una decisione nella stessa materia di poco più di un anno prima, dichiarava la necessità della separazione della telefonia fissa da quella mobile. Una separazione, lo ripeto, che contraddice l'opposta decisione assunta soltanto un anno e mezzo fa, quando venne dichiarata pubblicamente l'importanza strategica delle sinergie tra i due tipi di telefonia. Ci troviamo di fronte ad un' azienda il cui indebitamento pesa nella catena alta del controllo, cosa che come tutti sanno rende molto più complicata la riduzione del debito e molto più costose tutte le operazioni tese a tale riduzione. La Telecom, signor Presidente, ha 90.000 dipendenti; negli ultimi cinque anni ha dismesso tutti i suoi cespiti più preziosi, le società controllate che operano nel mondo, in Europa e fuori d'Europa, e il suo patrimonio immobiliare.

catena che detiene una partecipazione limitata e che pertanto non può permettersi di vederla ulteriormente diluita. Ebbene, davanti ad una situazione di questa gravità, davanti al pericolo di una crisi molto consistente della più grande azienda di telecomunicazioni del nostro Paese, noi impegniamo il Parlamento a discutere di una questione

scritto da una persona perbene che ha ritenuto - per senso di responsabilità - di doversi dimettere per averlo redatto e averlo inviato alla società Telecom. E oggi impegniamo il Parlamento a discutere di questo aspetto della questione e non del cuore del problema, ossia la crisi di una società decisiva per il futuro del nostro Paese. Credo che avremo nel futuro la possibilità di parlarne ancora e mi auguro che in quelle circostanze si metta a fuoco la questione principale a cui il Parlamento, la politica, il Governo debbono prestare l'attenzione. Signor Presidente, ho ascoltato le sue comunicazioni in apertura di seduta e mi è parso di sentire che saranno i Presidenti di Camera e Senato a decidere quale dei due rami del Parlamento vedrà il dibattito sulla questione sulla quale il Presidente del Consiglio ha dichiarato di voler venire a riferire. Non mi sembra che sia il Presidente del Consiglio a decidere in quale ramo del Parlamento verrà ma, se non ho inteso male dalle sue parole, saranno i Presidenti dei due rami del Parlamento a stabilire il calendario della discussione.

a favore del calendario e mi auguro che anche su questa decisione, in spirito di collaborazione,

Presidente, intanto vorrei tranquillizzare il collega Zanda: siamo noi dell'opposizione che chiediamo alla maggioranza di ripensare la votazione sul calendario Non abbiamo nessun motivo per votarlo, per una ragione molto politica: stiamo discutendo un calendario, signor Presidente, che tace sul solo punto politico che sta a cuore a tutti noi. Il fatto che si stia parlando della questione Telecom in sede di votazione del calendario in fondo dimostra che può essere persino l'unico momento nel quale il Senato della Repubblica si possa occupare di questo problema. il resto, sta alla disponibilità del Presidente del Consiglio decidere dove e quando andare il 28 - ci auguriamo che non abbia altri impegni quel e poi tendiamo a temere che scelga la Camera dei deputati. Non è un problema di gelosia di una Camera rispetto all'altra; piuttosto è la questione emersa con molta forza nel corso di questi dieci giorni da quando è cominciata la vicenda Telecom. Il Presidente del Consiglio non aveva alcuna intenzione di venire in Parlamento. La domanda è: perché dopo dieci giorni è stato costretto a dire sì? sì? Se avesse detto sin dal primo giorno che sarebbe venuto il 28 si sarebbe impostata in modo diverso la polemica con il Presidente del Consiglio e avremmo preso atto del fatto che riteneva normale, come gli era stato suggerito dall'amico, ex presidente della Camera, Casini, non considerare cosa da matti venire in Parlamento! La sua reazione è stata nelle prime 24 ore di dire che nulla sapeva! Addirittura ha detto: «Sono sorpreso che Telecom abbia questo progetto». Sembrava caduto dalle nuvole il Presidente del Consiglio per ricordare dieci giorni - non sono dieci mesi - la vicenda. Immediatamente dopo ha detto: «È da matti andare in Parlamento! Non ci vado!». E si è discusso in Parlamento cosa sarebbe dovuto avvenire. Da parte della maggioranza si è teso a dire: purché venga il Governo! Si è cominciato a parlare di Ministri competenti: abbiamo cercato di dire che il ministro di settore, lo sventurato onorevole Gentiloni, forse competente in materia di telecomunicazioni, era certamente ignorante sul punto specifico. Quindi, avremmo avuto in Parlamento un ministro ignorante della questione. La maggioranza ha detto: va bene. Fino a stamattina sembrava del tutto normale che venisse Gentiloni. La questione politica è: perché oggi il Presidente del Consiglio è stato indotto a dire sì? Solo perché una parte della sua maggioranza, della sua maggioranza, non dell'opposizione, lo ha indotto a fare una cosa doverosa. Allora la ragione è questa. Qual è la parte di questa maggioranza che si è spinta di più a chiedere questo, e perché lo ha fatto, e perché Prodi alla fine ha dovuto accettare? Non vi è dubbio che vi è stata una parte della maggioranza che ha ripetutamente affermato, anche con dichiarazioni pubbliche, anche nella Conferenza dei Capigruppo del Senato, che era opportuno che il Presidente del Consiglio venisse in Parlamento. Ecco la questione politica di fronte alla quale ci troviamo. Stiamo discutendo un calendario nel quale il rapporto tra la maggioranza e il Presidente del Consiglio chiude il rapporto Parlamento-Governo. Ecco perché l'opposizione, che aveva chiesto fin dall'inizio che il Presidente venisse a riferire in Parlamento, non è stata soddisfatta per oltre dieci giorni e oggi, improvvisamente, dopo la Conferenza dei Capigruppo della Camera - che, come sappiamo, non delibera il calendario, dà un orientamento politico - il Presidente del Consiglio è stato indotto a decidere in tal senso. È una questione sulla quale il Presidente del Consiglio deve riferire, è bene che glielo si dica, signor Presidente del Senato. Noi non siamo interessati a sapere se lui sapeva del documento Rovati o no, può continuare a mentire, è chiaro che nessuno gli crederà se dirà che non sapeva nulla. *(Applausi dal* Dobbiamo chiedere al Presidente del Consiglio - lo chiediamo fin d'ora - perché ha deciso di venire in Parlamento dopo che per dieci giorni ha detto di no, perché una parte della sua maggioranza lo ha spinto a dire sì; sì; evidentemente, ha messo in discussione proprio il rapporto tra Prodi e Rovati, proprio il rapporto tra Prodi e il suo consigliere economico. Questo problema è stato il motivo di una rottura del rapporto di fiducia tra il Presidente del Consiglio e una parte della sua maggioranza: di ciò occorre discutere.

non ha nessun interesse a discutere del caso Telecom come fatto politico generale, anche se all'interno della maggioranza di Governo vi sono componenti politiche interessate a capire se vi sono privatizzazioni sbagliate, da rivedere o meno. Questo è un problema che una parte del centro-sinistra intende discutere, e fa bene a forse non ne potrà discutere al Senato; pazienza! Questa è la ragione per la quale l'opposizione chiedeva che il Presidente del Consiglio intervenisse subito; abbiamo appreso che tornerà in Italia giovedì prossimo alle ore 12. Poteva venire giovedì pomeriggio, venerdì, sabato o domenica, poteva dare immediatamente una risposta positiva alla richiesta politicamente urgente dell'opposizione. Ha ritenuto di dire no all'opposizione ed è ovvio che l'opposizione non ha motivo di accettare un calendario rispetto al quale il Presidente del Consiglio dice di no; una parte della maggioranza lo approva perché ha ottenuto quello che voleva, cioè mettere a nudo cioè mettere a nudo le questioni politiche sulle quali il Presidente del Consiglio teneva chiuso nel suo rapporto con Rovati il problema del rapporto con la grande impresa Telecom. Questo è il problema che è esploso all'interno della maggioranza; per la prima volta, da maggio ad oggi,

di poter decidere da solo tu e il tuo consulente su tali questioni, perché sono questioni che ci riguardano tutti». Questo è il problema politico, signor Presidente. *(Applausi dal Gruppo UDC).* La maggioranza potrà ovviamente ottenere di non discutere del merito della questione, farà finta di discutere, come ha detto il collega Zanda, dei problemi di questa grande azienda,

Casualmente, come si è notato, proprio Guido Rossi, l'esperto in calcio negli stinchi, che è stato richiamato, prima dal calcio e ora dalla politica, perché la sua esperienza di calcio serve anche a questo.

Questa, collega Finocchiaro, era la problematica costituzionale posta nella Conferenza dei Capigruppo. Non c'è stata una collegialità del Consiglio dei ministri, non dico dei venti Ministri, ma neanche dei Ministri che rappresentano i partiti maggiori della maggioranza di Governo. Governo. La questione che è davanti a voi riguarda il Partito democratico, riguarda questa maggioranza e il rapporto con Prodi. Prodi tende al potere assoluto del Presidente del Consiglio, mentre una parte della sua maggioranza glielo nega. Questa è la questione aperta,

politiche della Telecom e su quanto avvenuto in questi anni e a ripensare insieme alla dialettica pubblico-privato, riformulando insieme una valutazione per cui nella vita economica non esiste il pubblico e il privato, ma aziende che funzionano e aziende che non funzionano, bene, la Democrazia Cristiana avrebbe tolto tanto di cappello a questa provocazione, anzitutto culturale, del Presidente del Consiglio. Non dimentichiamo infatti che, pur nella miseria elettorale in cui siamo precipitati, il partito storico al quale facciamo riferimento ha alle spalle le idee dei Fanfani, dei La Pira, di coloro che hanno ideato l'approccio cristiano all'idea di un'impresa pubblica. Non abbiamo quindi dogmi a discutere anche nel merito le provocazioni che abbiamo ascoltato poco fa in quest'Aula e che potevano venire dal Presidente del Consiglio: in tale caso, sì,

è un signore che ha rinunciato all'indennità, grande o piccola, che Palazzo Chigi poteva dargli; è un signore che si è assunto, anche in questa occasione, responsabilità superiori alle sue,

che non ci sia bisogno di appellarsi alla cavalleria per ricordare cosa accade nella vita delle aziende e nella vita politica. Io ho diretto alcuni giornali e quando un giudice scriveva

si trova di fronte a un collaboratore che ha sbagliato. Quando un Presidente del Consiglio ha un collaboratore che ha compiuto un atto su cui si è acceso il dibattito politico egli si presenta alla Camera o al Senato, in sala stampa, dove gli pare, ma ne risponde lui, se è il capo del Governo,

distacco lo rispediamo al mittente perché il piatto è gradito ma la testa non è quella giusta! Il Presidente del Consiglio, a fronte della crisi Telecom, tace

che, a furia di frequentare la Cina, egli abbia perso la strada della ragione politica seria che la vita democratica esige e che Capo di Governo che è al centro di un caso che accende l'attenzione del Paese e che riguarda un'azienda che ha 90.000 dipendenti, 5.000 dei quali già rimandati a casa per effetto della precedente privatizzazione,

ma naturalmente eserciteremo i nostri diritti e i doveri democratici di controllo in forme accettabili e democratiche, ma purtroppo sicuramente alternative a quella che avevamo sollecitato, che prevedeva un immediato e civile confronto in quest'Aula.

Mentre noi siamo riuniti a discutere dell'ordine dei lavori, i sindacati che rappresentano tutti i lavoratori della Telecom hanno proclamato uno sciopero generale per il 3 ottobre. La situazione del gruppo è talmente grave - 41 miliardi di *deficit*, se non sbaglio, quindi più della finanziaria che consideriamo già assai cara

con un'aggiunta, però, che la rende ancora più preoccupante: in questo caso, si tratta di uno dei settori strategici del Paese, perché l'informatizzazione coprirà tutti i settori, compreso quello della sicurezza, dunque sono questioni molto delicate. non sono d'accordo con la piega che ha preso questo dibattito, come ho detto oggi ai colleghi Capigruppo; non sono d'accordo perché credo che sia necessario un salto di qualità. Non possiamo continuare ad attardarci

intende fare una politica strumentale scandalistica, con un ruolo dell'opposizione in un certo modo e quello della maggioranza in un altro? Il Capo del Governo ha dichiarato che non era al corrente del piano. Io gli credo, ma gli credo anche perché, tutto sommato, quello che mi interesserebbe discutere è quando faremo il punto sul fallimento della politica delle privatizzazioni, chiunque le senatore D'Onofrio). So bene com'è andata la vicenda Telecom ma c'è un fallimento della politica delle privatizzazioni di cui, indipendentemente da come siamo collocati, dovremo prendere atto, prima o poi. La parte che rappresenta il Paese, quindi i lavoratori, e quindi i risparmiatori e il mondo produttivo, dovrà discutere di queste materie oppure Cosa ci può interessare sapere se il dottor Rovati era in buona fede o in malafede? È un piccolo scandaletto rispetto alle proporzioni della partita Telecom.

se riusciremo ad evitare che di fronte ai problemi del Paese si parli sempre di altro, se riusciremo a riportare il dibattito del Senato sulle questioni concrete, sull'ordinamento giudiziario, sulle Commissioni da varare, alcune delle quali di grande importanza, credo che avremo fatto qualcosa che il Paese potrà apprezzare. Non apprezzerà sicuramente una tensione nel Parlamento o in una Camera che impedisca di affrontare i problemi quotidiani e concreti delle persone.

Il senatore Schifani ha proposto di utilizzare la seduta di giovedì pomeriggio per un dibattito sulla vicenda Telecom poi auspicato che, magari solo come ascoltatore, il Presidente del Consiglio, che dovrebbe essere rientrato dagli Stati Uniti, sia presente. La seconda proposta è quella del senatore Castelli, che chiede (l'abbiamo ricevuta oggi e io l'ho vista) di mettere in calendario, se non sbaglio subito (ma "subito" bisogna vedere cosa vuol dire), la mozione relativa alla vicenda del discorso del Papa a Ratisbona.

due. Dovremmo ora procedere alla votazione di queste due richieste di modifica del calendario che prima vi ho illustrato. Se non ci sono obiezioni (io le ho richiamate tutte e due) e se il senatore Castelli ritiene di dover votare la sua proposta e non ritenesse

il mondo della giustizia presenta, mai come in questo periodo, notevoli complessità e sempre più spinosi problemi, alcuni, per la verità, non recentissimi che le varie strategie di intervento non sono riuscite a risolvere. Ai problemi della resa di giustizia, dell'arretratezza dell'apparato e della riorganizzazione degli uffici, si sono aggiunti quelli dell'ordinamento giudiziario, cioè di un sistema che un illustre giurista definì «il reticolo normativo dello statuto funzionale dei magistrati, importante quanto i codici e senza il quale gli stessi codici di rito non possono funzionare».

Sull'attività giudiziaria e sulla magistratura i Costituenti dettarono ben precise disposizioni rivolte a garantire l'esercizio della giurisdizione ad opera di un corpo giudiziario di alta professionalità, dotato al tempo stesso di autonomia e di indipendenza, nella VII disposizione transitoria previdero una nuova legge sull'ordinamento giudiziario formulata in piena conformità con la Costituzione. Ma l'ordinamento Grandi del 1941 ha continuato ad applicarsi, anche con successive modifiche ed integrazioni, e ciò ha suscitato nella letteratura giuridica una vasta elaborazione e sempre un vivace dibattito. Sono stati per la verità molteplici i tentativi di una riforma organica rimasti senza esito, sia per vedute ideologiche divergenti, sia per le difficoltà insite nei problemi stessi, anche perché le linee di fondo tracciate dalla Costituzione si pongono a mezza strada tra l'impianto francese del funzionariato della giustizia ed il sistema anglosassone del potere terzo. Dunque, un dibattito fervido ed agitato che dura però da 50 anni, troppi. E devo dare atto al senatore Castelli ed alla sua ex maggioranza di avervi posto mano, seppure a colpi di spada che per certi aspetti hanno inciso su quella indipendenza e su quella autonomia fermamente volute dalla Costituzione: colpi di spada che, che, come ben sappiamo, determinarono i messaggi correttivi del presidente Ciampi. La riforma però non ha segnato soltanto un ritorno in alcuni punti al sistema impiegatizio dell'ordinamento Grandi, sminuendo, tra l'altro, la centralità del Consiglio superiore della magistratura quale organo di governo dell'ordine giudiziario; ha anche determinato incidenze negative sullo stesso esercizio della giurisdizione per almeno due motivi: innanzitutto, perché oggi il problema di maggior rilievo, come si sa, questo modo lumacoso della giustizia di procedere, problema che la riforma dell'ordinamento non risolve affatto; in secondo luogo, perché alcune delle metodologie introdotte dalla riforma, come i concorsi per la progressione in carriera, distolgono necessariamente il giudice dall'attività quotidiana e lo spingono ad un carrierismo poco conforme all'esigenza di continuità e di impegno per una giustizia sollecita secondo i reali bisogni dei cittadini. Insomma, la riforma introdotta con la legge delega del 2005 e con i decreti attuativi, invece di riportare serenità (il che è giusto) ed ordine nel metodo della giustizia, ha accentuato contrasti e lacerazioni; per di più, in alcuni suoi aspetti rischia di rompersi alla prova dei fatti sul terreno della concreta operatività. Non intendo proporre, onorevoli senatori, una controriforma, né una riforma completamente diversa. Intendo piuttosto, con disponibilità personale e politica e con buon senso pratico, ricalibrare alcuni dei meccanismi posti dai decreti legislativi; per la verità, ad alcuni mi sono già applicato non cambiandoli assolutamente, registrandone però, rispetto a questa mia disponibilità a questo modo di rivisitare tratti dell'ordinamento, gli snodi per aggiustare quelle previsioni normative imprecise, contraddittorie o pericolose per l'autonomia della magistratura. Con il disegno di legge in esame ho soltanto chiesto la sospensione dell'applicazione di alcuni decreti legislativi riguardanti la riforma dell'ordinamento giudiziario ed ho ritenuto di farlo sia per evitare alla macchina giudiziaria, già abbastanza disastrata, ulteriori incidenze negative, sia per la necessità di elaborazione ed approvazione di provvedimenti correttivi. Nessuna lesa maestà, quindi, rispetto ai provvedimenti posti in essere precedentemente, né la voglia matta di una contrarietà in via di principio. Al riguardo, faccio rilevare che proprio qualche giorno fa il vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura, già autorevole componente di questa Assemblea, senatore Mancino, con l'equilibrio e la saggezza che caratterizzano la sua grande esperienza istituzionale, ha sottolineato come il Consiglio corra il rischio di operare nella costante incertezza e di avviarsi verso una vera e propria paralisi di alcuni dei settori di governo della magistratura, soprattutto - ha detto il presidente Mancino - in quello disciplinare. Ha espresso così il senatore Mancino l'auspicio che l'istituzione consiliare possa contare su un solido e permanente tessuto normativo che non determini anomalie nel governo dell'ordine né di trattamenti differenziati nell'esercizio di tale governo. È rilevante, fra l'altro, che da nessuna, dico nessuna, delle componenti consiliari, pur rappresentanti appezzamenti di territorio politico espresse da quest'Aula e dall'Aula della Camera, si sia levata una qualche voce di dissenso sulle preoccupazioni espresse dal senatore Mancino. E le sue parole di buon senso le ho considerate non, come ha forzatamente detto qualcuno, un'indebita incursione nei lavori parlamentari, assolutamente no, ma come la fotografia realistica di un disagio, la constatazione di un'emergenza censita da parte sua e sottoposta alla nostra attenzione con spirito sereno e sgombro da pregiudizi. Io l'ho letta così e mi piace leggerla così. È dunque indispensabile e urgente che il Parlamento adotti le sue determinazioni sulla mia proposta di rinviare di alcuni mesi l'entrata in vigore dei decreti di riforma, cioè per il tempo strettamente necessario a correggere quelle anomalie che incidono negativamente sullo *status* dei magistrati, ma, quel che più conta e m'interessa di più, sull'efficienza della giurisdizione. In qualcuno, lo so, fa capolino l'idea che, mandata in esilio questa riforma, non si arriverà mai più ad altra riforma e ad altra conclusione operativa, finendo così quasi in una critica terra di nessuno, in una sorta di indistinto costituzionale senza alcun approdo finale. Non sarà così, non è questa la mia intenzione e garantisco la mia parte politica e il Governo che non sarà così. Da collega con una qualche esperienza parlamentare comprendo la legittima esigenza espressa dalle opposizioni di sapere cosa c'è a ridosso della sospensiva, cioè quali innovazioni intende con me il Governo proporre a modifica della riforma Castelli. Si tratta, riconosco, di un'esigenza legittima, che ho già cercato (ma, mi rendo conto, invano) di soddisfare con le mie comunicazione alle Commissioni giustizia di Camera e Senato, in questa occasione voglio però, con maggior dettaglio, con una fotografia meno panoramica e più scattata appunto nell'indagine della vicenda giudiziaria, dar conto a quest'Assemblea del lavoro di revisione dei decreti legislativi, un lavoro pressoché ultimato a livello propositivo. Voglio anche chiarire che il programma futuro non potrà consistere, non è mia intenzione farlo consistere, nel ripristino della situazione esistente prima dell'attuale ordinamento. Non invoco, né spero, né lavoro per un semplice ritorno al passato. Dico subito allora che le innovazioni non toccano i decreti legislativi nn. 20, 24 e 35 del 2006, concernenti taluni incarichi direttivi di legittimità, l'organico dei giudici addetti alla Cassazione e la pubblicità degli incarichi extragiudiziari, il cui contenuto, senatore Castelli, mi trova concorde. Dico pure che le modifiche non soltanto rispondono al criterio dell'essenzialità perché toccano punti di assoluta importanza, ma non contraddicono ai criteri ispiratori della riforma rivolti ad assicurare la massima serietà per l'accesso in magistratura, la costante professionalità dei magistrati e il relativo controllo da parte degli organi di governo dell'ordine giudiziario, la unitarietà dell'ufficio di procura, l'attribuzione di funzioni sulla base delle attitudini specifiche, il necessario rigore nel regime disciplinare. Qual è allora, da parte mia, il tentativo difficile, complicato, qual è il filo esile di Arianna per riuscire a determinare una possibilità di cittadinanza alle idee che in questo momento sto trascrivendo e ponendo alla vostra attenzione? Ecco il contenuto delle possibili innovazioni, cominciando dal concorso in magistratura fino al sistema disciplinare. Per l'accesso in magistratura, dirò per quelli più addetti e più dotti anche di me in materia, ritengo si debba conservare quell'impronta di concorso di secondo grado verso cui già si orientava la riforma Castelli con il decreto legislativo n. 160 del 2006; anzi l'ho maggiormente, dal mio punto di vista, caratterizzata nei presupposti di ammissibilità e nelle prove. Propongo infatti alla vostra attenzione che possano partecipare alle prove non i semplici laureati in legge, ma coloro che abbiano già superato un concorso pubblico, o che siano docenti in materie giuridiche con due anni di anzianità, ovvero iscritti all'albo degli avvocati da almeno due anni; il presupposto può anche consistere nell'aver completato il primo incarico di giudice onorario con conferma, oppure nell'aver svolto le funzioni di deputato, senatore, consigliere regionale, provinciale o comunale; al di fuori di questi casi, condizione essenziale è il diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali. Un'eccezione si può fare e credo sia giusto farla per quei giovani che, laureatisi con voto altissimo e con un *curriculum* di tutto rispetto, potrebbero essere costretti a rinunziare al concorso perché la condizione della loro famiglia non consente consistenti attese. Mi sembra opportuno, inoltre, che alle tre prove scritte ne sia aggiunta una quarta, a carattere pratico, consistente nella redazione di una sentenza; ciò consente di accertare la padronanza delle tecniche argomentative, la sensibilità ad una congrua ed equilibrata motivazione e la capacità di qualificare la situazione concreta nell'astratta fattispecie normativa che il semplice elaborato a tema assai spesso non esprime. L'originario testo sull'accesso obbliga gli aspiranti ad una scelta iniziale tra l'esercizio delle funzioni giudicanti e requirenti. A parte - debbo dire, onorevoli senatori - le critiche suscitate nella cultura giuridica e nel mondo giudiziario, alcune concrete considerazioni mi hanno indotto a proporre l'abolizione di quest'obbligo iniziale: in primo luogo, chi intende partecipare al concorso, specie se ha il solo titolo di specializzazione, non ha consapevolezza piena delle funzioni esercitabili e quindi non è in grado di operare un'opzione che potrebbe durare per l'intera carriera; c'è infine l'esigenza degli uffici, che incide notevolmente sulla distribuzione funzionale, mentre le scelte iniziali rischiano di sottrarre agli organi di governo della giurisdizione la politica del personale, con possibili e gravi discrasie tra settore giudicante e settore requirente.

la definizione anticipata dei criteri per la valutazione omogenea degli elaborati, la distinzione in gruppi di lavoro, nella prospettiva di accelerare l'*iter*, in modo che si possa rispettare la cadenza annuale dei concorsi. Come si vede, all'accesso si vorrebbe dare un'impronta di notevole serietà, anche in linea con talune esperienze straniere, in maniera particolare quelle europee; e analoga serietà al tirocinio iniziale, che si prevede sia curato da un intero settore della scuola della magistratura, con una organizzazione esclusivamente finalizzata al tirocinio. L'istituzione della scuola superiore della magistratura è una aspirazione da tempo avvertita dalla magistratura e dalla cultura giuridica: do atto con compiacimento a chi l'ha proposta di averla finalmente istituita. Le modifiche che propongo al riguardo sono poche e attengono soprattutto alla funzionalità operativa (e sottolineo funzionalità operativa) con alcune semplificazioni organizzative ed anche con sensibilità per gli impegni economici. In sostanza, le proposte di modifiche accentuano l'autonomia scientifica, didattica e gestionale della scuola, ne caratterizzano meglio i settori di intervento, con riguardo alla preparazione dei magistrati di prima nomina, alla formazione permanente attraverso *stage* periodici o di riqualificazione, alla cultura, molto importante, questa sì manageriale, degli aspiranti dirigenti di ufficio. La partecipazione del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero al direttivo della scuola è su base paritetica, oltre il prezioso apporto dell'avvocatura e dell'università. Scarse e, per così dire, non di rilievo ideologico sono le modifiche proposte in relazione al decreto legislativo n. 25 del 2006, concernente i consigli giudiziari e l'istituzione del consiglio direttivo della Cassazione: si tratta, onorevoli senatori, di puntualizzazioni in ordine al coordinamento normativo e di qualche correzione di semplice dettaglio. Più incisive, invece, sono le modifiche che si potrebbero apportare al decreto legislativo n. 160 del 2006, in tema di progressione di carriera; ciò perché al sistema dei concorsi interni per accedere a gradi superiori e a funzioni più alte, dei quali lo stesso decreto n. 160 fa una minuziosa e - diciamo la verità - anche un po' farraginosa classificazione, intenderei, con il consenso del Parlamento, sostituire il più incisivo sistema della verifica quadriennale concernente la capacità, la diligenza, la laboriosità e l'impegno. Come già dissi alle Commissioni giustizia, le leggi sui ruoli aperti non hanno dato buona prova di sé, e la mia proposta ne abbandona il criterio di fondo, così come fa la riforma Castelli. Ma il sistema concorsuale del citato a parte lo stigma impiegatizio che sembra riprodurre l'ordinamento del 1941, pone questi interrogativi rimasti senza risposta: quante volte e per quanto tempo ogni magistrato si sottrarrà all'ordinario esercizio della sua attività per dedicarsi alla preparazione dei vari concorsi interni? Come potrà non distrarre il suo impegno dalla giurisdizione? Quale stimolo ad un carrierismo indifferente alle sorti della giustizia questo sistema inocula nell'ordine giudiziario? In sostanza, la possibilità di partecipare ai concorsi, con la prospettiva di vantaggi di carriera e i relativi risvolti economici, potrebbe indurre molti a scegliere questa strada, abbandonando quegli uffici di primo grado dove si adottano le decisioni con maggiore impatto, soprattutto di natura sociale. Tutto ciò in contrasto con l'interesse del cittadino ad avere un magistrato esperto fin dal primo grado del processo. Viceversa, le valutazioni periodiche a tempi ravvicinati possono costituire non solo il presupposto per altre funzioni, ma anche importanti momenti di verifica, suscettibili di concludersi, se di esito negativo, con il blocco della progressione economica o con la destinazione ad altra funzione di chi si riveli inidoneo, addirittura, io ritengo, con la rimozione dei magistrati che non superino successive valutazioni. Tali verifiche potrebbero articolarsi, oltre che nell'autorelazione dei magistrati, sui rapporti dei capi degli uffici, sul riscontro di produttività, sui corsi di aggiornamento presso la scuola della magistratura, su segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati per fatti incidenti sulla professionalità o su specifiche situazioni di non indipendente esercizio della funzione ovvero, in conclusione, su comportamenti sintomatici di mancanza di equilibrio. Insomma, si tratta a questo punto anche di definire una sorta di banca dei dati valutativi da utilizzare per tramutamenti e per funzioni cosiddette superiori, per incarichi semidirettivi e direttivi; nulla impedisce comunque di attivarla in riferimento a situazioni comunque relative alla capacità, come ho detto, laboriosità, professionalità specifica, all'equilibrio e alle attitudini del magistrato. Quanto alle funzioni di legittimità, va in primo luogo garantito che, in linea con la Costituzione, il sistema resti nell'ambito della competenza del Consiglio superiore. Tuttavia il Consiglio ben potrebbe avvalersi di un apposito gruppo di magistrati e professori universitari per una prima valutazione dei provvedimenti degli aspiranti finalizzata al riscontro delle specifiche attitudini. Insomma, per l'accesso alle funzioni di legittimità la prospettiva è certamente diversa: un magistrato, per quanto bravo nell'attività di merito, può non essere in grado di svolgere una funzione di legittimità e perciò l'aspirante deve saper dimostrare la capacità di analisi delle norme. Tutto questo non può non essere integrato con la partecipazione ad appositi *stage* presso la scuola, che vanno frequentati da quanti aspirino a funzioni diverse. Su questi presupposti di controllata idoneità, secondo l'esito positivo della seconda e rispettivamente terza o quarta o quinta valutazione di professionalità, e sulla base di rigorose procedure concorsuali per titoli nonché di partecipazione a specifici corsi, si potrebbe fondare anche il delicato sistema degli incarichi semidirettivi, direttivi ed apicali; in proposito si deve tener conto delle specifiche attitudini organizzative, di gestione e della capacità di rapporto con il personale e l'utenza - la scuola ha in proposito uno specifico settore di formazione - nella prospettiva, sottesa all'articolo 107 della Costituzione, di porre l'uomo giusto al posto giusto; peraltro intenderei confermare la temporaneità di tali incarichi con rinnovi molto circoscritti e previo giudizio di idoneità. Vengo alla questione del passaggio dalla requirente alla giudicante e viceversa. Intenderei, sempre con l'assenso e il volere della maggioranza - che spero sarà ampia - di quest'Aula, conservare appieno il principio della distinzione delle funzioni affermato nella riforma Castelli: il passaggio è consentito a seguito della frequenza di un corso di qualificazione professionale, è subordinato ad un giudizio di idoneità specifica per il quale è possibile acquisire il parere del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ma il passaggio non è possibile in una sede compresa nel medesimo distretto; l'unica eccezione si potrebbe prevedere per il magistrato che abbia avuto una prima assegnazione, cioè dopo il tirocinio iniziale, per il quale l'incompatibilità è nell'ambito del circondario e non del distretto. Le modifiche, quindi, che intendo apportare al decreto legislativo n. 106 relativo all'ufficio di procura conservano appieno quel carattere unitario dell'ufficio del pubblico ministero che la riforma Castelli ha ribadito. Il capo della procura rimane nella piena titolarità dell'ufficio e dell'azione penale; a lui competono l'organizzazione e gli indirizzi della politica giudiziaria, l'assegnazione dei procedimenti, la determinazione dei criteri generali cui il sostituto deve attenersi, lo specifico assenso in tema di custodia cautelare e di sequestri, nonché i rapporti con i *media*. Insomma, non intendo affatto contrastare la necessità di ridisciplinare la procura secondo un modello diverso dagli uffici della giudicante, così da restituire ai procuratori quella unitarietà di indirizzo, che intemperanze e deviazioni purtroppo riscontrate nella prassi hanno talvolta annullato; tuttavia non è possibile, anche per motivi di funzionalità, stringere l'attività dei sostituti in un letto di Procuste ove scompare ogni e pur limitata autonomia, ove è mortificata la dignità professionale ed è stimolata una mentalità burocratico-impiegatizia per cui conta solo ciò che vuole e decide il capo e soltanto il capo. Nel contempo, attribuire tutta la responsabilità dell'intero ufficio al solo procuratore può determinare l'ingestibilità della procura, soprattutto di medio-grandi dimensioni, deresponsabilizza gli altri magistrati perché li pone al riparo di eventuali contestazioni disciplinari essendo il capo l'unico responsabile sia *in* *eligendo*, per la scelta dei sostituti assegnatari, sia *in* *vigilando*, per il *deficit* di controllo e il mancato esercizio del potere di revoca; né sarebbe facile per il CSM trovare magistrati disposti ad assumersi un peso tanto grave. Per queste considerazioni credo di poter proporre circoscritte modifiche, e cioè: come è stato chiesto da molti, ad esempio dal senatore D'Onofrio, la trasmissione al CSM dei criteri generali dettati dal procuratore per settori di indagine, affinché il consiglio possa fare le sue valutazioni; l'«assegnazione» e non la semplice «delega» ai sostituti, assegnazione che, conferendo facoltà operative con limitata autonomia funzionale, risulta responsabilizzante e coerente a quel principio della sottoposizione «soltanto» alla legge che secondo la Corte costituzionale vale anche per i magistrati del pubblico ministero; ovviamente la gestione del procedimento va pur sempre realizzata secondo i criteri generali dettati dal procuratore ed è revocabile motivatamente, con un controllo da parte del Consiglio superiore su richiesta del sostituto; l'eliminazione di addendi terminologici che, senza alcun apporto di qualificazione tecnica, caricano di valenze verticistiche ed assolutistiche un apparato della giurisdizione e attribuiscono ingestibili e totalizzanti responsabilità al solo procuratore. D'altronde, l'effettività e l'ampiezza dei suoi poteri restano integre nonostante le modifiche proposte; infine una più razionale disciplina della posizione dei procuratori aggiunti e del vicario, in un quadro più razionale di gestione dell'ufficio. Al sistema disciplinare è dedicato il decreto legislativo n. 109 del 2006 che introduce due innovazioni di base, cioè la tipicizzazione degli illeciti e l'obbligatorietà dell'azione disciplinare: le condivido entrambe, onorevoli senatori, per cui anche qui a mio parere le modifiche proposte sono abbastanza circoscritte rispetto all'impianto generale della riforma precedente. Quanto alla tipicizzazione, alcune formule risultano impraticabili o incomplete oppure equivoche o contraddittorie. Faccio qualche esempio. La formula adottata per il difetto di motivazione come illecito disciplinare rischia di imporre in ogni caso inutili e defatiganti spiegazioni in fatto per provvedimenti seriali o privi di rilevanza, come, ad esempio, le archiviazioni; la formula relativa all'omissione di rapporto si riferisce ai presidenti di sezione e di collegio ma trascura i procuratori aggiunti; l'espressione «comportamento reiterato» - richiamato dall'ordinamento giudiziario Castelli - è più precisa e stringente dell'altra «comportamento abituale». Vorrei eliminare, inoltre, laddove fosse possibile, alcune anomalie che si riscontrano in tema di illeciti da condotte estranee all'esercizio delle funzioni; così, ad esempio, l'espressione «condotta tale da compromettere l'immagine del magistrato» risulta esteriore e semplicemente formale, mentre è preferibile riferirsi alla «credibilità del magistrato»; in tema di divieto di iscrizione a partiti politici - divieto, onorevoli senatori del centro-destra, che rimane la previsione, come illecito, del «coinvolgimento in attività di centri politici» è troppo generica e può comprendere anche manifestazioni culturali senza alcun radicamento partitico, perciò suscettibile di incidere su diritti di libertà costituzionalmente garantiti. Ci sono infine formule come «l'uso strumentale della qualità» e «ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza e l'imparzialità», che risultano assolutamente incompatibili con la tipicizzazione e finiscono per attribuire la determinazione della condotta illecita ai titolari dell'azione o all'organo disciplinare. decreto n. 109 trasforma in obbligatoria l'azione disciplinare del procuratore generale; questa obbligatorietà, accompagnata dal dovere di rapporto a sua volta sanzionato, sta già determinando un enorme aggravio - di questo ha parlato il senatore e in seguito lo determinerà per la sezione disciplinare, rischiando di lasciare impuniti, anche per effetto della riduzione a metà dei termini di prescrizione, casi certamente meritevoli di essere perseguiti. Ad evitare questa conseguenza, proporrei due innovazioni. La prima riguarda il recupero di una disposizione che, opportunamente inserita nello schema originario, fu poi eliminata, e che consiste nella «non configurabilità dell'illecito disciplinare quando la condotta non incide negativamente, in concreto, sulla credibilità, sul prestigio o sul decoro del magistrato o sul prestigio dell'istituzione giudiziaria», cioè sui valori fondamentali oggetto di tutela; la seconda riguarda invece l'attribuzione al procuratore generale presso la Cassazione del potere di archiviazione quando la condotta non è disciplinarmente rilevante o non rientra in nessuna delle ipotesi tipiche oppure non è commessa con dolo o colpa grave o quando è già intervenuta la prescrizione. esprimo per la verità forti dubbi su quella figura del delegato del Ministro (e parlo di un delegato che potrei eventualmente delegare se fosse in atto questa riforma) inserito nel procedimento disciplinare che può esaminare testimoni, consulenti, periti e interrogare l'incolpato: si tratta di una figura anomala che sembra avere il compito di controllare lo stesso rappresentante dell'accusa, creandosi una marcata e irragionevole disparità nella simmetria «accusa-difesa» nonché possibili e preoccupanti situazioni di contrasto tra il procuratore generale e il rappresentante del Ministro circa la gestione processuale. In conclusione, onorevoli senatori, non si tratta, come ho letto anche oggi in questo frasario, in questo lessico, per chi ha motivato e poteva motivare diversamente o esprimersi in contrarietà con il mio provvedimento, di un'altra riforma, non si tratta di assumere soltanto elementi di discontinuità, né si tratta di un'iniziativa volta a indebolire l'orditura ordinamentale a tutto vantaggio della magistratura.

uno che riesce a tenersi in equilibrio, in questo caso propenda, anche con la sua stazza e con il suo peso, dalla parte della magistratura e non abbia un senso di equilibrio; in realtà esso rimane immutato, perché questo è lo stile e questa è la componente - non accessoria, ma importante - della mia vita politica e parlamentare.

altre, le più numerose, attengono a profili di impraticabilità delle norme o sono dirette ad evitare effetti di ricaduta assolutamente negativi per lo stesso governo del corpo giudiziario, mettendo in crisi, come ho detto, la stessa attività del Consiglio superiore. superiore. La sospensione, onorevoli senatori, è dunque necessaria e urgente per operare gli aggiustamenti descritti e per evitare che nel frattempo discrasie e anomalie normative ricadano sull'efficacia del senso di giustizia a cui dobbiamo applicarci, cioè su quel valore essenziale con cui ogni riforma deve necessariamente misurarsi. è di ostacolo all'intervento sospensivo il fatto che gran parte dei decreti sia già vigente. Alla sospensione, di per sé non in contrasto con i princìpi generali, il legislatore ha più volte fatto ricorso in occasione di riforme importanti, anche di natura ordinamentale; cito tre casi: l'istituzione del giudice di pace è stata ripetutamente differita e la seconda volta con un provvedimento adottato nove mesi dopo che quelle norme avevano acquistato efficacia; la nuova disciplina relativa alla segreteria e all'ufficio studi del CSM è stata differita fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e la norma di differimento è stata emanata ben cinque anni dopo la vigenza dell'originaria disciplina; l'entrata in vigore della normativa in tema di efficacia delle sentenze straniere è stata rinviata con un provvedimento legislativo adottato oltre un anno dopo l'efficacia di quelle riforme. Ricordo infine che la sospensione proposta sarà accompagnata da disposizioni transitorie per fare salvi gli effetti già prodottisi durante la vigenza dei decreti legislativi. Comunque, onorevoli senatori, onorevoli colleghi, a prescindere dalle posizioni che saranno assunte - tutte legittime - dai vari Gruppi parlamentari, continuo e continuerò a ritenere e sono convinto più che mai che bisognerà assieme (e sottolineo assieme), maggioranza e opposizione, lavorare allo e sullo stesso telaio istituzionale della giustizia. Anzi, a questo proposito si potrebbe - perché no - studiare una sorta di comitato ristretto che abbia a collaborare con il Governo e che metta appunto e a ruolo questa significativa e obbligata partecipazione di tutti per rendere omogenei i criteri che dovranno ispirare, secondo una corretta visione di intese istituzionali, il nuovo ordinamento giudiziario. Credo che questa sia una questione, la giustizia, che è elemento da intesa istituzionale perché su questi temi è giusto che ci sia la misura e il senso delle istituzioni, che tocca tutte le parti in causa presenti in quest'Aula. Occorre mettere allora a punto un nuovo contenitore il più possibile condiviso. Questa è la mia intenzione e i prossimi mesi ci diranno quali tessuti usciranno da quel telaio. Le riforme a mio parere intanto incidono e hanno un seguito nella coscienza popolare e hanno un esito favorevole nella pubblica opinione se partono da un confronto tra le forze politiche e se questo confronto è assunto come dato permanente, non come momento di episodicità. Un confronto che auspico, onorevoli senatori, né compiacente, né populista, ma che sappia riflettere anche - perché no - le ragionevoli esigenze dei destinatari dei provvedimenti che si vanno ad assumere. Le riforme non si possono fare sulla testa e totalmente contro chi, poi, le deve attuare. Una coalizione politica, a qualunque schieramento appartenga, non può non tener conto di questo elementare criterio di buon senso politico. In conclusione, credo che se ci imporremo tutti una serena valutazione sul come disegnare un nuovo modello ordinamentale, privi dello stress politico che assai spesso frequentiamo, se tutti considereremo le riforme, e questa riforma in particolare, non come uno sfondamento di linea contro gli altri, allora il risultato sarà di qualità e avremo contribuito, ognuno per la sua parte, a ricercare le misure più adatte, perché al centro della giustizia italiana, sempre più europea, ci sia finalmente solo e soltanto il cittadino come arbitro.

seguire il discorso del ministro Mastella per il frastuono che c'era in Aula, a testimonianza dell'assoluto disinteresse

Questo è il dato fondamentale sul quale dobbiamo ragionare: qual è la vera materia del contendere di questo provvedimento? Ciò che è scritto nelle leggi? No,

deve legiferare la magistratura o il Parlamento? Questo è il problema fondamentale che noi siamo chiamati a dirimere in questi giorni.

che è sotto gli occhi di tutti: ha aperto il Ministero all'ANM e ha detto: prego, il Ministero è qui, lottizzatevi le posizioni apicali, basta che non mi date problemi. Anche plasticamente, vediamo seduto ai banchi del Governo un magistrato, che è stato preso direttamente dal tribunale e portato qui a rappresentazione plastica e anche formale di quanto conti la magistratura sugli altri poteri dello Stato in questo momento. Quindi, da un lato vi è la magistratura al Governo e in Parlamento

questo è il dato di fatto. L'ha ripetuto lei perché la questione dei controlli più stringenti è un cavallo di battaglia dell'Associazione nazionale magistrati. Qual è Qual è il problema fondamentale e inaccettabile in questo momento per la magistratura? Si dice che il giudice è autonomo e indipendente, ma il giudice non è mai stato meno autonomo e indipendente come in questo momento: il giudice è completamente nelle mani del Consiglio superiore della magistratura, che a sua volta è nelle mani dell'Associazione nazionale magistrati e delle correnti, questo è il dato fondamentale.

se non gestisci la magistratura secondo i voleri dell'Associazione nazionale magistrati, devi andare via! Il caso Cordova *docet*. Cordova era un uomo di destra? No! Era semplicemente un uomo che non intendeva soggiacere ai *diktat* dell'ANM ed è stato cacciato via dal Consiglio superiore della magistratura, gestito dalle correnti. Questi sono i punti fondamentali che stasera dobbiamo dirimere. Inoltre lei, mi scusi, ministro Mastella, ha fatto anche un po' di confusione, perché da un lato ci ha fatto alcune proposte sui decreti legislativi che oggi sono in esame, ma ci ha anche parlato della scuola della magistratura che intende modificare. Guardi che non è in esame questo provvedimento, lei non ha proposto la sospensione di questo decreto legislativo,

lei ha dimostrato, attraverso le sue proposizioni, che sarebbe possibile seguire questa strada, anche più ragionevole, e cioè lasciare che la legge esplichi i suoi effetti

È ovvio: nessuno pretende di aver fatto una legge perfetta. È chiaro che una riforma così complessa avrà dei buchi, avrà dei problemi e quindi andrà corretta, è stato previsto nella legge.

«Castelli *delendum* *est*», questo è il punto fondamentale. Il Ministro che ha osato varare una riforma contro il parere della magistratura va cancellato, la riforma va cancellata come elemento plastico per definire il potere della magistratura in materia di giustizia. Questo è il punto fondamentale su cui dobbiamo ragionare. Dunque va cancellata la riforma, perché nessuno crede che si tratti soltanto di una sospensione: questa è un'eutanasia!

che non possiamo accontentarci e non ci accontentiamo delle sue proposizioni su questo punto. Una posizione seria potrebbe essere quella di metterci intorno a un tavolo con il Governo che ci dica quali sono i reali effetti negativi che questa riforma ha portato, perché nessuno fino a questo momento, e neanche il Ministro stasera, ci ha riportato un solo

la maggioranza di Governo intende procedere ad una riforma istituzionale come quella che riguarda i rapporti con la magistratura anche tenendo conto dell'opposizione oppure Ritiene di essere autosufficiente nei rapporti con la magistratura oppure no? Questa è la questione che abbiamo posto. Vogliamo sapere se c'è volontà di procedere d'intesa con l'opposizione. Ovviamente, l'opposizione, che era maggioranza nel precedente Parlamento, ha prodotto una riforma legislativa e accetta di tutto ragionevole buon grado le modifiche da apportare, dicendosi pronta a votarle anche immediatamente, in modo che non ci sia più alcun bisogno di sospendere il provvedimento. Se invece ci si dice: «Prima sospendete e poi campa cavallo...», ovviamente non crediamo che il cavallo campi. Occorre essere molto precisi su questo punto. sono un testardo: ho motivo di ritenere che tra oggi e la settimana prossima, quando dovremo votare questo provvedimento, il Governo possa maturare un orientamento diverso di fronte alla nostra dichiarata disponibilità a votare immediatamente (lo ripeto) le modifiche

nella sua comunicazione non ha più parlato di sospensione del provvedimento, ma ha fatto riferimento a norme transitorie sulle quali si dovrebbe intervenire per ragioni di funzionalità. Non ha più parlato, il senatore Mancino, in qualità di Vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, di sospensione del provvedimento. Questo è un fatto istituzionale di enorme rilievo,

Siamo pronti in questo momento a modificare l'ordinamento vigente per evitare disfunzioni istituzionali, ma non riteniamo necessaria alcuna sospensione del provvedimento adottato anche perché non vorremmo, onestamente, essere presi in giro. Si definisce sospensione quella che di fatto è un'abrogazione.

Modifichiamo l'ordinamento vigente, dimostriamo che cerchiamo l'intesa istituzionale di tutto il Parlamento con l'ordine giudiziario. Se questa è la volontà siamo pronti, se questa non è la volontà siamo costretti a ritenere preferibile mantenere il provvedimento così

Signor Presidente, abbiamo ascoltato con attenzione l'intervento del ministro Mastella ed ora i due interventi dei colleghi Castelli e D'Onofrio. La mia opinione è che nel discorso del ministro Mastella vi siano, in un'esposizione analitica che potrà essere forse apprezzata meglio leggendo il testo, le linee direttrici di un intervento modificativo delle norme dei decreti delegati della cosiddetta legge Castelli che può realizzarsi per venire incontro a problemi e obiezioni che da più parti sono state avanzate. Il ministro Mastella ha più volte sottolineato che la volontà del Governo non è quella di abrogare una parte delle norme esistenti, perché abrogazione significa esclusivamente cancellazione,

nuova legge sull'ordinamento giudiziario approvata nella scorsa legislatura. E' evidente che la prima questione posta dal collega D'Onofrio trova già risposta

legge Castelli, ma che deve essere definita in un confronto e in una convergenza con le forze dell'opposizione. l'esigenza di interventi modificativi non nasce da un ragionamento astratto e da una scelta ideologica, ma da un'analisi concreta delle inadeguatezze delle norme attualmente vigenti. La mia proposta è che nella situazione attuale, avendo di fronte a noi una proposta del Governo (e devo credere che il disegno di legge

a partire dal Senato, cioè dal ramo del Parlamento davanti al quale il ministro Mastella ha enunciato le linee guida degli interventi modificativi da apportare alla cosiddetta legge Castelli.

ritengo che noi dobbiamo, senza drammatizzare e senza attribuire un particolare significato politico a questa scelta, fermare per un momento l'applicazione e l'entrata in vigore effettiva

fermare una parte dei decreti ma, nel momento stesso in cui stiamo discutendo della proroga, bisogna avviare il lavoro sul merito degli interventi modificativi, bisogna costituire e far funzionare un Comitato ristretto. Chiediamo al Governo che la sua proposta venga depositata in questi giorni e che su di essa si possa avviare un lavoro nel merito. Mi sembra che questo sia un possibile punto di compromesso.

consentire un lavoro comune in un Comitato ristretto ed anche il varo di norme che trovino un consenso quanto più possibile ampio. A tale riguardo, chiedo un gesto di buona volontà al senatore D'Onofrio e agli altri colleghi. Se fosse possibile accordarci su questo punto, massimo sarà l'impegno del Gruppo dell'Ulivo, in Comitato ristretto e in Commissione, per farsi carico delle ragioni che verranno avanzate dall'opposizione e per fare presto a giungere a norme che risolvano i problemi che sono sul tappeto e che ci trovino, quanto più possibile, d'accordo.

la Commissione affari costituzionali non ha potuto esprimere il parere su questo disegno di legge per mancanza di numeri nella maggioranza. Il parere,

colleghi e riconosciuto dal Ministro, i tre decreti legislativi dei quali si chiede la sospensione sono già entrati pienamente in vigore:

nel testo giunto in Commissione propone che questi tre decreti legislativi vengano sospesi, ancorché abbiano dispiegato i loro effetti. Nulla si dice sulla disciplina che sarà applicata a decorrere dal giorno della sospensione, né sulla disciplina intercorrente tra il giorno della sospensione e il giorno dell'entrata in vigore. Presidente, noi stiamo facendo un'operazione legislativa. L'Aula rischia di mandare in porto un'operazione legislativa che non ha precedenti. Si tratta di un salto nel buio, di una vergogna giuridica, di un obbrobrio parlamentare. Non è mai capitato nella storia del Parlamento - e credo non si trovino precedenti negli annali giuridici - che una legge già modificata nel suo cuore e abrogata totalmente, in maniera implicita o espressa, riviva grazie alla sospensione della legge che ne ha provocato l'abrogazione. si tratti di una situazione unica nel panorama legislativo. Purtroppo, non è la prima stranezza di questa legislatura. Vorrei far presente tra l'altro, signor Presidente, che vi sono materie estremamente sensibili toccate da questi decreti legislativi. è la materia del disciplinare, per cui ove non si ponesse mano a risolvere questa grave lacuna, che riguarda sia il futuro successivo alla sospensione, sia il periodo intercorrente tra la sospensione e e l'entrata in vigore di questi decreti legislativi che si vorrebbe sospendere, si verificherebbero problemi gravissimi, perché avremmo comportamenti di magistrati, degli uffici di tutti coloro che sono soggetti a queste norme che non ricadrebbero né nell'una, né nell'altra disciplina. Un vero obbrobrio giuridico. che a questa situazione possa porre rimedio la proposta emendativa del Governo, che si è accorto con qualche mese di ritardo

decidessimo una sospensione degli effetti del codice penale Rocco e stabilissimo che nel frattempo si attuano gli effetti del codice penale precedente. Non vi è alcuna differenza di carattere formale tra queste due ipotesi, ma credo che l'esempio possa servire a capire l'enormità di una simile questione. Presidente, signor Ministro, è una questione che tocca non una materia ordinamentale di carattere secondario,

di legge e che quindi non può essere sostituito da norme di altra natura; è un ordinamento che ha una rilevanza costituzionale e sul quale abbiamo sul quale abbiamo realizzato un grande progetto di riforma, ancorché nel 1948 la nostra Carta costituzionale prevedesse l'attuazione in poco tempo della riforma dell'ordinamento giudiziario.

senatore Pastore e dal senatore Castelli. Questa mi sembra la decisione che l'Aula potrebbe adottare e che,

finestra") *(Ulivo)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ritengo che la questione pregiudiziale sia completamente destituita di ogni fondamento. Sono anzi convinto che il suo accoglimento presenterebbe problemi e dubbi più consistenti sotto il profilo della legittimità costituzionale. Già in altra sede l'attuale vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, l'onorevole Mancino, ha avuto occasione di segnalare i danni anche gravi all'attività del Consiglio superiore della magistratura e degli uffici giudiziari stessi determinati dall'entrata in vigore e dall'efficacia dei tre decreti che ci riguardano. Ha usato anche toni piuttosto pesanti parlando di situazioni di blocco o di rischio di blocco dell'attività e anche di situazioni di caos. Ritengo che l'entrata in vigore di questi tre decreti legislativi in particolare si presenti in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione che è quello che tutela il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, ma ci sono altri profili di dubbio di legittimità costituzionale più consistenti. I primi riguardano il decreto legislativo n. 106 del 2006 relativo alla gerarchizzazione delle procure della Repubblica. Le critiche di maggior rilievo vengono rivolte in particolare modo nei confronti di questo decreto legislativo perché inficia gravemente il principio costituzionale dell'indipendenza della magistratura, in particolare nell'articolo 104 della Costituzione, che fa riferimento alla magistratura come ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. all'articolo 109 che dice che l'autorità giudiziaria dispone direttamente, come autorità giudiziaria e quindi come potere diffuso, della polizia giudiziaria. Ricordo

proprio impedendo un capillare e diffuso esercizio dell'azione penale che si va ad inficiare la natura stessa di questo potere diffuso.

e, in particolare, alla tipizzazione - verso la quale peraltro non siamo contrari - e alla obbligatorietà dell'azione disciplinare in ogni caso. È strettamente collegata, come complessità e come rischio di danno, questa entrata in vigore con quello che dicevo in materia di indipendenza e autonomia della magistratura, in riferimento all'esercizio del potere del pubblico ministero. L'azione disciplinare, così com'è stata prospettata e così com'è entrata in vigore, crea dei problemi particolari all'interno del Consiglio stesso, rischiando di creare, contrariamente a quanto viene detto, un blocco dell'attività disciplinare dell'attività disciplinare per il Consiglio superiore della magistratura; d'altronde, proprio per il numero eccessivo di azioni, di segnalazioni e di esposti nei confronti di magistrati nei confronti di magistrati si creerebbe da una parte il blocco degli organi che sono stati istituzionalmente incaricati di questa azione disciplinare e, dall'altra, questo carico il raggiungimento in tempi brevissimi del termine della prescrizione, che sappiamo essere fissato in un anno. Quindi, da una parte la moltiplicazione incontrollabile del numero dei procedimenti (con effetti

è persino lapalissiano ricordare come la previsione, così com'è stata fatta, di concorsi ripetuti per i magistrati (il problema della progressione in carriera) costringerebbe i singoli magistrati a pensare più ai concorsi che non all'attività giudiziaria con dispendio di energie e di tempo in attività extragiudiziali e contro quel principio di natura costituzionale - che ricordavo all'inizio del mio intervento - relativo al buon andamento della pubblica amministrazione. L'unico problema serio che poteva e che potrebbe sorgere è relativo al periodo transitorio, così com'è stato segnalato dall'intervento del senatore Pastore; periodo transitorio è stato individuato correttamente ed esattamente dall'intervento del Ministro. In particolare, il Governo ha presentato un emendamento

La seconda parte di questo articolo 4-*bis* fa riferimento, ancora una volta, agli effetti che si sono prodotti e alle situazioni che si sono esaurite nel vigore dei decreti legislativi

del Senato, ci sono proposte anche dell'Ulivo che riguardano proprio la modifica della normativa in tema di ordinamento giudiziario, con particolare riferimento ai tre decreti legislativi che sono oggetto di discussione questa sera. Si diceva che non si vuole abrogare, si vuole correggere. È una mano tesa questa; si vuole arrivare tutti assieme alla correzione dei punti negativi che sicuramente esistono, come peraltro diciamo che alcuni punti positivi esistono. Questi vanno recuperati e, laddove c'è la necessità,

approvata la proposta del disegno di legge del Governo.